"Il link apre una nuova finestra"). L'elenco dei senatori in congedo e assenti per incarico ricevuto dal Senato, nonché ulteriori comunicazioni all'Assemblea saranno pubblicati nell'allegato B al Resoconto della seduta odierna.

Onorevoli colleghe e colleghi, prima di dare inizio ai nostri lavori sono certa di rappresentare il comune sentimento di solidarietà della nostra Assemblea alle popolazioni dei centri delle Marche e dell'Umbria, che ieri sera e stanotte sono state colpite da violente scosse di terremoto. L'epicentro del sisma si è registrato nel maceratese e ha colpito principalmente i paesi di Visso, Ussita, Castelsantangelo sul Nera e Preci, dove si registrano gravi danni alle strutture abitative e ai monumenti storici, artistici e religiosi. Ancora una volta, dopo soli due mesi dalla terribile notte del 24 agosto, il Paese è in ansia per la sorte di territori già duramente messi alla prova da eventi calamitosi. Rivolgiamo un sentito ringraziamento alle donne e agli uomini impegnati nella macchina dei soccorsi, che si è immediatamente mobilitata per assistere le popolazioni coinvolte, alle quali il Senato della Repubblica rinnova sinceri sentimenti di vicinanza e, ancora, di solidarietà alle persone che stanotte hanno dovuto dormire fuori casa. *(Applausi).* L'ordine del giorno reca la discussione del disegno Signora Presidente, oggi è il 27 ottobre 2016,

A una mia precisa richiesta in Commissione, la risposta è stata puntuale: a tutt'oggi il Governo non ha presentato alle Camere il disegno di legge di stabilità. Che il Governo non osservi una legge non è propriamente educativo, se così si può dire. Ma la gravità sta nel fatto che l'Unione europea, con una lettera di ieri o di avantieri, si è pronunciata sul Documento programmatico di bilancio e si sofferma su alcune grandezze che coinvolgono l'elemento fondamentale della legge di stabilità, cioè i saldi di finanza pubblica. Il Governo, sempre per via giornalistica, dice, parlando di un documento che noi non conosciamo, che la manovra rimane così com'è, ma non giustifica, né può farlo perché non esiste il documento che va giustificato. Siamo in una situazione, signora Presidente, imbarazzante sul piano istituzionale. Le chiedo di rappresentare al Presidente del Senato di richiamare immediatamente il Governo alla presentazione della legge di stabilità. Questo è un episodio senza precedenti. Signora Presidente, non è un problema dell'altra Camera, bensì di questa Camera insieme all'altra. Il Presidente del Senato ha titolo, anzi legittimazione, a richiedere che immediatamente il Governo presenti alle Camere la legge di stabilità o, ove decida di modificare qualcosa sulla base della lettera dell'Unione europea, di farlo adeguandolo con una nuova Nota di aggiornamento al DEF. Peraltro, una nuova Nota di aggiornamento già avrebbe dovuto essere fatta, perché l'ufficio parlamentare del bilancio, nella nota successiva successiva alla presentazione del documento di bilancio, ha detto che la manovra è diversa nella composizione e c'è una norma che prescrive che, quando una manovra è diversa nella composizione, deve essere riproposta al Parlamento perché dobbiamo conoscerla.

non saremmo in grado, ove mai ci fossero state delle audizioni, di poter parlare di qualsiasi elemento relativo alla legge di stabilità. Pertanto le chiedo, signora Presidente, di interessare immediatamente il Presidente per svolgere questo atto: è un presidio

colleghi, prima di entrare nel merito dell'illustrazione mi permetta di unirmi alle sue parole. Svolgo questa relazione con il pensiero fisso

con la convinzione che quelle popolazioni e quei territori sapranno superare un'altra prova così difficile. È stato grazie alla solidarietà e alla prontezza delle istituzioni che in questi due mesi disperazione e paura non hanno vinto e, invece, ha vinto la volontà di riscatto, che anche questa volta vincerà, di quelle popolazioni e quei territori. Vengo, signora Presidente, al disegno di legge che è oggi oggetto di esame, già approvato alla Camera, che reca la ratifica dell'accordo di Parigi

La necessità di ridurre le emissioni è quanto mai urgente. Il 2016 è considerato da molti scienziati l'anno più caldo e inquinato mai vissuto dal nostro pianeta, da quando esistono rilevazioni, con concentrazioni *record* di anidride carbonica; è una situazione di grande allarme, stigmatizzata dal recente rapporto redatto dall'organizzazione meteorologica mondiale. Secondo questo documento, tra il 1990 e il 2015 si è registrato un aumento del 37 per cento dell'effetto radiante dei gas ad effetto serra, rimasti troppo a lungo nella nostra atmosfera: anidride carbonica, metano, protossido di azoto, prodotti

(400 parti per milione), destinate a rimanere tali per molti decenni e quindi a pesare non solo su di noi, ma soprattutto sulle generazioni future. È quindi necessario un intervento urgente le misure contenute nell'accordo oggi al nostro esame vanno nella giusta direzione. L'accordo è stato sottoscritto, voglio ricordarlo, da 191 Paesi, quindi dalla quasi totalità di quelli esistenti, già ratificato da 86 Stati, tra cui Stati Uniti, Cina, Brasile, India, oltre a oltre a molti Stati europei. Entrerà in vigore il prossimo 4 novembre, a meno di dodici mesi dalla sua stipula, un tempo insolitamente breve per accordi di questo tipo.

aveva impiegato oltre otto anni per entrare in vigore. Sarebbe un segnale molto importante se l'Italia potesse concludere il procedimento di ratifica in tempi brevi questo è l'obiettivo odierno - per arrivare alla prima riunione della Conferenza delle parti, prevista a Marrakech per il prossimo 7 novembre, con la ratifica avvenuta. Si tratta peraltro di un testo ampiamente condiviso, L'accordo di Parigi è destinato a sostituire l'impianto dell'attuale Protocollo di Kyoto e fissa una serie di impegni giuridicamente vincolanti, che sono ambiziosi ma al tempo stesso realistici per le parti contraenti, stabiliti in base ai diversi contesti nazionali. L'obiettivo di lungo periodo è quello di limitare l'aumento della temperatura al di sotto dei due gradi centigradi rispetto ai livelli preindustriali, con l'intento di continuare gli sforzi

cambiamenti climatici non sono solamente di carattere ambientale: drammatici flussi migratori che coinvolgono diverse parti del mondo sono per tanta parte provocati proprio dai cambiamenti climatici. Il riscaldamento globale provoca siccità, desertificazione, uragani ed è, dunque, un potentissimo fattore di spinta dei flussi migratori, in particolare da alcune regioni africane. In relazione all'obiettivo di riduzione degli effetti dei cambiamenti climatici, ogni Paese, stando a questo trattato, è tenuto a redigere e a comunicare, al momento della ratifica, la sequenza dei contributi nazionali per la mitigazione A differenza del Protocollo di Kyoto, l'Accordo di Parigi non presenta un annesso vincolante in cui siano definiti gli obblighi di riduzione dei gas per le parti, proprio in ragione del fatto che i contributi vengono determinati a livello nazionale in autonomia, fermo restando il loro carattere vincolante una volta notificati. Segnalo che l'Unione europea e i suoi Stati membri sono stati tra i primi a indicare il proprio obiettivo, che è la riduzione delle emissioni di almeno il 40 per cento entro il 2030. Il trattato rappresenta un punto di svolta e incoraggia le parti a compiere sforzi per conservare e migliorare i bacini di assorbimento di gas ad effetto serra e, in particolare, dell'anidride carbonica, il cui incremento è strettamente connesso ai cambiamenti climatici. Il trattato, altresì, incoraggia le parti a investire risorse economiche contro gli effetti negativi delle emissioni che derivano soprattutto dalla deforestazione. Un altro degli obiettivi fondamentali dell'Accordo è favorire una trasformazione delle economie, rendendo nel lungo periodo tutti i flussi finanziari compatibili con l'impegno di riduzione delle emissioni ad effetto serra, prevedendo da parte dei Paesi più ricchi un impegno finanziario, trasparente e monitorato, a sostegno dei Paesi in via di sviluppo. Rientrano in questo obiettivo il trasferimento di tecnologie e l'accrescimento delle capacità organizzative di questi Paesi, nonché il sostegno a politiche di educazione ambientale e civica per una maggiore trasparenza delle informazioni in materia. Viene anche previsto un meccanismo di monitoraggio delle emissioni, con l'impegno per le parti di riferire e sottoporre alla verifica multilaterale i progressi nell'attuazione dei rispettivi piani, per tracciare un avanzamento verso gli obiettivi collettivi

dal 7 al 18 novembre (sarà la COP22). A tale organismo partecipano non solo i Paesi contraenti, ma anche le organizzazioni regionali di integrazione economica, a partire quindi dall'Unione europea, nei settori di loro competenza. Voglio ricordare che la Conferenza di Marrakech sarà chiamata a discutere

una risoluzione che stimola un impegno ancora maggiore degli Stati membri; il Consiglio dell'ambiente ha approvato un documento, anche con punti critici, sui preparativi della Conferenza di Marrakech il Comitato europeo delle Regioni, signor Presidente, ha formulato a sua volta una serie di indicazioni, sottolineando, tra l'altro, l'importanza delle Regioni e degli enti territoriali, accanto agli Stati nazionali, nel raggiungimento degli obiettivi di riduzione delle emissioni. L'accordo di Parigi infatti - e anche questo è un aspetto da sottolineare positivamente - ricorda che l'impegno di riduzione dei cambiamenti climatici non può essere assolto dai soli Stati centrali, che pure sono le parti firmatarie, ma necessita del coinvolgimento attivo degli enti sub-statali, delle città, dei privati e delle società territoriali, delle imprese e dei cittadini. In conclusione, Presidente, voglio ricordare che il disegno di legge di ratifica si compone di 6 articoli. Gli articoli 1, 2 e 6 riguardano rispettivamente l'autorizzazione alla ratifica, l'ordine di esecuzione e l'entrata in vigore. L'articolo 3 è invece dedicato al finanziamento del fondo internazionale sul clima, istituito nel 2010 durante la sedicesima sessione della Conferenza delle Parti della Convenzione Si tratta del principale strumento finanziario della Convenzione, che ha, dunque, un ruolo centrale nel convogliare risorse per le politiche di attuazione degli impegni assunti a livello internazionale. Questo disegno di legge autorizza il Ministro dell'ambiente ad assicurare la partecipazione italiana a tale fondo, con una spesa di 50 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2016 al 2018, per contribuire alla prima capitalizzazione. L'articolo 4 stabilisce che eventuali contributi nazionali, che fossero definiti a livello europeo, vengano autorizzati con provvedimenti normativi *ad hoc*. L'articolo 5, infine, riguarda la copertura del provvedimento. Gli oneri collegati direttamente alla ratifica e all'esecuzione dell'Accordo sono quantificati in circa 490.000 annui per le spese di missione, a partire dal 2017, cui vanno aggiunte ulteriori spese pari a 1,450 milioni di euro per il 2017 e a 2 milioni circa a Signor Presidente, varare l'Accordo di Parigi, farlo entrare in vigore al più presto, riempirlo di contenuti ulteriori significa riappropriarsi di una fortissima volontà volontà politica, per essere finalmente protagonisti nell'affrontare uno dei temi più drammatici che riguardano noi e, soprattutto, le generazioni a venire, verso le quali abbiamo l'obbligo di lasciare un pianeta in salute.

la sfida fondamentale del XXI secolo - ha detto qualche anno fa Jeffrey Sachs - sarà prendere atto che l'umanità condivide un destino comune in un pianeta affollato. Il destino comune che ci attende porta con sé la responsabilità di agire per tutelare il pianeta, cioè la nostra vita. Una responsabilità che è emersa chiara dalle parole dei *leader* riuniti a Parigi lo scorso anno per COP21, dove ho avuto l'onore di essere capo delegazione per il Parlamento italiano. Nell'aprire la Conferenza di Parigi, che ha portato a sottoscrivere l'accordo che oggi siamo chiamati a ratificare in via definitiva, il segretario generale Ban Ki-Moon ha ricordato che è l'ultima possibilità per salvare il clima, un'occasione unica che potrebbe non tornare. il presidente Obama ha aggiunto che siamo la prima generazione a subire l'impatto dei cambiamenti climatici e l'ultima a poter fare qualcosa. Questa consapevolezza e questa responsabilità - questa presa d'atto, per restare alle parole di Sachs - sono finalmente largamente diffuse, tanto da aver coinvolto a Parigi 193 Paesi, responsabili del 96 per cento delle emissioni. L'Italia è arrivata a Parigi tra i pochi Paesi ad aver rispettato gli impegni di Kyoto: dal 1990 abbiamo ridotto le nostre emissioni del 23 per cento e produciamo da fonti rinnovabili un terzo dell'energia consumata. Importante è stato inoltre il contributo della Presidenza italiana dell'UE alla costruzione dell'avanzata posizione europea, come importante è stato il nostro ruolo nello sciogliere i punti di conflitto nella trattativa fatta fatta a Parigi, per cui ringraziamo il Ministro ancora oggi. Con la ratifica dell'accordo confermiamo il nostro impegno a lavorare per tenere l'innalzamento della temperatura sotto i due gradi, possibilmente fermandoci a 1,5 gradi. La ratifica, inoltre, ci permette di continuare a partecipare con protagonismo ai prossimi appuntamenti, a partire da COP22 che inizierà a Marrakech, come diceva il relatore, dal 7 novembre. Un protagonismo che deve essere nostro, certamente, ma ancor di più europeo. Veniva detto giustamente che l'Unione europea ha ratificato il 4 ottobre l'accordo di Parigi, ma già a marzo 2015 aveva condiviso un impegno a ridurre le emissioni di gas a effetto serra del 40 per cento rispetto al 1990. Dopo l'approvazione dell'Accordo da parte dell'Europa abbiamo anche raggiunto quel traguardo del 55 per cento dei Paesi firmatari che hanno ratificato che serviva per renderlo effettivo. Insomma, dal prossimo 5 novembre avremo in vigore un accordo storico, capace di unire tanti Paesi - dalle grandi potenze, a Stati piccolissimi - intorno a obiettivi vincolanti per tutti, ma - giustamente - con modalità di realizzazione degli impegni calati sulle caratteristiche di ciascun contesto nazionale e con un sistema condiviso di *governance* internazionale. Approvando il disegno di legge oggi in discussione e completando la ratifica dopo il voto della Camera dei deputati, diamo seguito anche noi agli impegni presi, stanziando le risorse necessarie per i progetti pilota, per informare ed educare e per contribuire al Green climate fund (il Fondo verde per il clima), per il quale lo stanziamento è di 50 milioni l'anno per il triennio 2016-2018.

un accordo che fosse stato calato dall'alto e avesse imposto a ciascun Paese le cose da fare avrebbe rischiato di essere un atto nobile, ma poco aderente alle necessità e alle scelte politiche di ciascun Governo. Lasciare a ciascun firmatario l'onere di autoimporsi vincoli stringenti è invece una scelta che mi pare ci aiuti a far crescere davvero la consapevolezza delle istituzioni e delle società e far essere l'Accordo davvero una scelta di ogni Paese. Le questioni climatiche - è bene che anche su questo si arrivi a una larga consapevolezza - rischiano non solo di danneggiare l'ambiente, ma anche di acuire disuguaglianze e produrre cambiamenti il cui impatto si annuncia davvero travolgente. Negli ultimi duecento anni (l'era definita Antropocene, nella quale per la prima volta l'uomo ha un impatto determinante sulla natura) l'impronta umana sulla terra è cresciuta enormemente, con la popolazione sestuplicata,

con un livello di inquinamento che ha alterato in maniera sostanziale gli equilibri del pianeta. Gli scenari per il 2100, senza interventi urgenti, decisi e concreti sono inquietanti: tra i tre e i sei gradi delle temperature medie, l'innalzamento di due metri del livello del mare, 200 milioni di possibili rifugiati climatici e un aumento del 50 per cento del fabbisogno energetico mondiale. La questione riguarda davvero tutti - i Paesi sviluppati, così come quelli in via di sviluppo - ed è evidente come le questioni ambientali siano strettamente connesse a quelle sociali ed economiche. Non possiamo più considerare l'ambiente in cui viviamo come qualcosa di particolare ed estraneo a noi, ma dobbiamo sempre più integrarlo in tutte le politiche: si tratta dello spazio in cui viviamo e nulla può prescindere da questo.

che rilanci gli obiettivi di uno sviluppo sostenibile, così come è stato fatto all'ONU nel settembre 2015, incoraggiando anche le imprese e sostenendole a puntare su fonti energetiche sostenibili, innovazione, nuove tecnologie, creatività e ricerca. tutti fattori presenti nel DNA dell'Italia, che dobbiamo saper riscoprire, valorizzare e modernizzare, ma - soprattutto - sostenere e incentivare. In questo senso, dobbiamo anche superare la storica contrapposizione tra obblighi ambientali e diritto allo sviluppo, trovando nuove forme di collaborazione tra Paesi e nel Paese, anche con quel meccanismo di differenziazione di oneri e obblighi e di scambio di conoscenze previsto dallo stesso Accordo di Parigi. Come sostiene l'ONU con l'Agenda 2030, lo sviluppo sostenibile riguarda tutti i Paesi e impegna tutti i Governi. L'obiettivo n. 13 dei 17 approvati nel settembre 2015 riguarda proprio il cambiamento climatico e la sfida a limitare l'aumento della temperatura e del suo impatto.

Lo sviluppo sostenibile, inteso in questo nuovo modo, è la cornice dentro il quale collocare ogni nostra scelta e ogni nostro agire per il futuro. È fondamentale che non sia soltanto - diciamo così Ecco perché il provvedimento che oggi siamo chiamati a votare è davvero così importante. Non possiamo però nasconderci: quello di oggi, colleghi, è soltanto un primo passo e anche dopo la ratifica definitiva dell'Accordo in esame dovremo continuare costantemente, seriamente e concretamente il nostro impegno. Serve guidare il mondo davvero verso una nuova fase. Serve che la politica si dimostri capace di leggere, interpretare e governare i cambiamenti, che ormai caratterizzano stabilmente la nostra società e i processi di trasformazione ambientale, demografica e industriale, che sono in atto e che non si fermeranno. Lo ripeto: lo dobbiamo almeno alle prossime generazioni, se non anche a noi stessi, che oggi siamo in vita. Serve una rivoluzione *green*, articolata in ogni settore, per cambiare in profondità gli stili di vita, rendere consapevoli le cittadine e i cittadini di quanto importante sia questa sfida e attivare tutte le istituzioni, ciascuna per le proprie specifiche responsabilità. Infine, questa scelta deve diventare politica *mainstream* del legislatore, guidando ogni scelta e ogni politica, come elementi di un complessivo e sostenibile impegno con il futuro di tutti. Per le donne e gli uomini il possibile precede il reale ed è questa capacità che oggi dobbiamo riscoprire, abbandonando il determinismo e riprendendo in mano il cambiamento, orientandolo al benessere e alla sostenibilità. È una sfida complessa ed epocale, rispetto alla quale, ratificando l'Accordo in esame, dimostriamo di essere pronti. Dal momento del voto in avanti, però, dovremo dimostrare anche di esserne concretamente all'altezza. *(Applausi

di sette anni saremo a 450 parti per milione. Ci saremo per forza, anche se adesso le emissioni di CO2 venissero stabilizzate. Quindi il livello di 450 parti per milioni per la sola CO2 è irrealizzabile:

Bisognerebbe conoscere la macchina termica planetaria. Io che mi diletto un po' di queste cose, giusto per farmi un'idea, ho osservato la mappa della nevosità sulla calotta glaciale groenlandese, che è uno dei punti più critici per il nostro sistema planetario non tanto per il livello il regime delle nevicate sulla calotta groenlandese è completamente cambiato. Laddove prima nevicava ad ovest, adesso nevica ad est, quindi abbiamo già una modifica della circolazione dei venti a livello dell'emisfero nord, e questa è una cosa assolutamente non prevista e non prevedibile. In secondo luogo, non conosciamo le dinamiche di riscaldamento e di raffreddamento superficiale degli oceani, non sappiamo perché il ciclo ENSO passi da positivo a negativo, non sappiamo perché si crei il "blob atlantico" atlantico" che determina il clima europeo. Non sappiamo molte cose e ci affidiamo a concetti come le teleconnessioni che sono legami probabilistici tra un evento che accade in una parte del mondo e un altro evento che avviene da un'altra parte del mondo. Tutte cose non studiate. In base a questo, noi pretendiamo di poter dire che un grado e mezzo sia una soglia di sicurezza, quando poi arrivano studi, uno dietro l'altro, che parlano della instabilizzazione di una parte della calotta antartica dovuta all'infiltrazione di acque calde. Quindi noi non possiamo stare tranquilli pensando che se sale la temperatura di un grado e mezzo va bene perché farà mediamente un grado e mezzo in più su tutto il pianeta

niente copertura ghiacciata significa assorbimento di maggiore calore dagli oceani. Noi non sappiamo bene come il calore oceanico venga distribuito. Conosciamo la circolazione termoalina,

inchioda al fatto di limitare le emissioni di CO2 ad un livello che è

le proiezioni dicono che saremo vicini alle mille parti per milione. Ma qualcuno potrebbe dire che non riesce a capire che cosa siano queste benedette mille parti per milione. Non lo riesce a capire nemmeno chi ha fatto il progetto EPICA (European project for ice coring in antartica), cioè una carota che arriva fino al fondo, al basamento della piattaforma continentale, nel tentativo di studiare come fosse la concentrazione atmosferica dei gas milioni di anni fa, quando ha cominciato a costituirsi la calotta antartica. Bene: le mille parti per milione non sono mai state

apparentemente io me ne posso fregare di un gas che è considerato inodore, incolore e non tossico, non posso fregarmene del fatto che la concentrazione di ossigeno atmosferica scende, perché è l'ossigeno quello che noi respiriamo. Ma supponiamo anche per un attimo che noi decarbonizzassimo adesso, con il nostro livello di 402 parti per milione di CO2 in atmosfera più tutti gli altri gas. Questo comporterebbe un altro effetto a catena che ancora non è stato compreso. Quello che è certo è che l'incremento medio di temperatura non si riflette in un incremento locale uguale. L'ho appena detto: in questo momento l'oceano artico misura anomalie positive di 15 gradi ma i dati dell'ultimo anno parlano di più 3,7 gradi sull'artico. La zona polare artica è quella più sensibile insieme con la zona circumartica. Nella zona circumartica ci sono enormi depositi di metano intrappolati. Sempre per chi non lo sapesse, il metano ha un GWP (*global warming potential*) di 35 volte, cioè una molecola 35 volte più grande di quello di una molecola di CO2 e le emissioni di metano sono quelle più legate alla destabilizzazione della tessitura dei terreni. Questa è un'altra delle cose che non è studiata, ma il principio di precauzione dice che se io non conosco è meglio che non vada a interferire.

dati storici che parlano di queste emissioni improvvise e incontrollate, sia dal fondo dell'oceano che dal terreno. L'evento di cinquanta milioni di anni fa nel Nord atlantico testimonia esattamente questo: metano intrappolato sotto il mare, a livello del basamento marino che si è improvvisato sviluppato nell'atmosfera.

quindi, può andare avanti anche senza di noi. Tutto ciò che stiamo dicendo lo stiamo dicendo solo a nostro uso e consumo. Ma qui delle due l'una: o decidiamo di riuscire a stare in pace con questo pianeta o decidiamo di non farlo. Questo accordo decide di non farlo, di ignorare il problema, chiudendolo dietro una parvenza di sicurezza. Ma ricordiamo che qui non c'è alcuna sicurezza e tutto diventa sempre un problema di denaro. Noi abbiamo addotto il problema economico come il primo motivo per non intervenire su questo. Eppure, ogni studio fatto ha testimoniato quanto segue: il denaro investito nella decarbonizzazione e nella rimozione frutta molto più profitto del denaro investito nella mitigazione o nel *business as usual*. Perché, alla fine, si parla di incremento delle energie rinnovabili ma mai di spegnimento delle centrali a fonti fossili; si parla sempre di economia additiva e mai di economia sottrattiva. Anche in questo caso, le parole sono importanti. Si parla di sviluppo sostenibile. Ma l'espressione sviluppo sostenibile è stata creata da chi ha creato l'eternit!

arriva dell'olio di palma perché l'Unione europea ha deciso che vuole attuare una strategia sui biocarburanti, che è una strategia che sta distruggendo l'agricoltura delle altre Nazioni, io dico no. Non voglio il biocarburante europeo e non mi piace come si sta procedendo. Se qualcuno vuole vendere in Italia del biocarburante fatto con olio di palma, in Germania, io impongo una tassazione tale per cui la vendita diventerà improponibile. Devo fare la scelta giusta. Poi la Germania si lamenterà? Che si lamenti pure. Noi siamo pur sempre la settima o l'ottava potenza economica al mondo e nessuno al mondo può permettersi di non commerciare con l'Italia. Noi abbiamo una potenza contrattuale che dobbiamo sfruttare. Non dobbiamo sempre andare al traino. Parliamo dell'Unione europea, che si è riempita la bocca parlando

Quindi, la *road map* dell'Unione europea è una *road map* del tipo: andiamo avanti così che ci arriviamo spontaneamente. Cosa non negata alla COP19 dalla stessa delegazione tedesca quando ci abbiamo parlato personalmente. Quindi, non sto dicendo cose inventate, ma cose che la delegazione tedesca ha detto in una riunione. Gli Stati Uniti hanno già raggiunto il loro picco e stanno diminuendo rispetto al loro picco, sempre per lo stesso motivo. Perché l'industria, spontaneamente, sta decarbonizzando per maggiore efficienza raggiunta. Quindi, questo accordo non fa altro che assecondare qualcosa che sta già avvenendo. Il caso cinese e quello indiano sono casi a parte, ma anche loro avranno lo stesso tipo di curva. Quello che noi non ci possiamo permettere è che tutti raggiungano il loro picco. Questo è scritto nell'accordo. È scritto che le Nazioni devono affrettarsi a raggiungere il picco. Non c'è scritto che non devono raggiungerlo o che devono averlo messo alle spalle. C'è scritto invece che devono affrettarsi a raggiungerlo e ciò vuol dire che si considera che le emissioni continueranno ad aumentare e sto parlando della sola CO2. Quindi, che aspetta il nostro Governo a impuntarsi in tutte le sedi internazionali e fare da apripista? Infatti, se decidessimo di mettere in campo strategie tecnologiche e fiscali per fare questo, il circuito virtuoso scatterebbe immediatamente. L'industria è molto più pronta dei politici che ci sono dietro, fino a che alla borsa elettrica il costo dell'energia è parametrato sul costo del produttore marginale, quello che fa l'energia con il carbone, non ne usciremo mai. Cosa aspettiamo a fare una mossa innovativa e mettere fuori legge le centrali a carbone? Non è difficile. Il carbone, essendo un prodotto vecchio di 300 milioni di anni, contiene al suo interno qualunque sostanza, comprese sostanze radioattive e metalli pesanti. Basta imporre una limitazione al camino e una centrale a carbone non ha più la possibilità di esercire. Non è difficile. Abbiamo bisogno di 5.000 megawatt a carbone? Non abbiamo bisogno di 5.000 megawatt a carbone, ma semplicemente

Tassiamo di più l'energia, prodotta con fonti fossili, che arriva dall'estero, allora: è giusto e sacrosanto che lo si faccia. Creiamo un fondo apposito con quella tassazione per continuare, non dico la decarbonizzazione, ma - vado oltre - l'estrazione.

praticamente le riserve di petrolio dell'Iran, il tutto per avere un parco mucche. Tutto questo si trasformerà in CO2. Quindi, di cosa stiamo parlando?

Ma finché la sola agricoltura emetterà circa 50 miliardi di metri cubi di metano, non andremo mai da nessuna parte. chiaro? Per cui, se non interveniamo su questo (che sono le cose più semplici), abbiamo finito. Le emissioni cumulate di CO2 e di metano del settore zootecnico cubano dal per cento delle emissioni globali di gas a effetto serra, più di tutte le centrali a carbone, più di tutte le automobili, gli aerei, le navi o qualunque altro veicolo mosso da un motore endotermico: tutti questi veicoli messi insieme fanno meno della semplice zootecnia. abbiamo il problema davanti agli occhi e lo ignoriamo. Sarebbe semplicissimo intervenire su questo: basterebbe che il Governo togliesse i sussidi. La carne, il latte e i derivati dovrebbero costare, come tutte le cose, il giusto; non un prezzo volutamente calmierato, perché questa si chiama distorsione del mercato. E se ancora il WTO non se ne è accorto, se ancora l'Unione europea non si è accorta che questi sono meccanismi distorsivi, bisogna che qualcuno li avverta. Vi sembra ragionevole che la carne abbia un costo comparabile a quello delle verdure? dei cereali? A me sembra che ci sia una leggera distorsione. Ma di quanti soldi stiamo parlando? La politica agricola comunitaria, come si continua a chiamare, è il capitolo di spesa più ricco dell'intera Unione europea: tutti i soldi veicolati per sostenere un settore che da solo non sta in piedi.

quando la macchina termica di un pianeta si inceppa e non si riesce più a tenerla sotto controllo. Sto parlando del pianeta Venere: questo pianeta ha trovato il suo equilibrio a circa 320 gradi, perché il calore intrappolato continua a restare intrappolato. Noi non dobbiamo e non possiamo permetterci di aspettare che il pianeta trovi un suo equilibrio, ma molto semplicemente perché una situazione può diventare irreversibile. Una volta che fosse andata in crisi la calotta artica o che fosse andato in crisi l'Antartide occidentale, quanto dovremmo aspettare perché il pianeta possa riprendersi? Dovremmo aspettare, come minimo, l'inizio di un nuovo periodo glaciale. Finché non si hanno le condizioni per ricreare quella struttura, anche se si decarbonizza e si torna a livello di 280 parti per milione (che sono quelle stabili dell'era preindustriale),

Salutiamo le studentesse e gli studenti dell'Istituto comprensivo «Valle dei Laghi» di Dro, in provincia di Trento. Diamo il benvenuto al Senato anche ai loro insegnanti.

rispetto alla ratifica di questo trattato che abbiamo giudicato importantissimo sin dall'inizio, sin da quando è cominciata la discussione. Lo abbiamo considerato, anche nelle versioni precedenti, come un impegno del nostro Paese nostro Paese assolutamente da rispettare ed, anzi, da sostenere per quanto sia, come si è già detto, sempre insufficiente rispetto agli obiettivi che ci dobbiamo porre di risanamento ambientale del nostro pianeta.

già previsto: ciò rischiava di lasciarci in una veste di osservatori di fronte alla comunità internazionale. Una comunità internazionale che, come abbiamo detto da sempre, deve essere più sensibile a questi temi. L'abbiamo detto perché riteniamo che la questione ambientale sia una questione di questi tempi e di queste ore. L'abbiamo detto anche perché la questione ambientale porta con sé grandi problematiche di natura sociale;

di coloro che vogliono approfittare di tutto senza alcun rispetto dei parametri di vita dell'insieme. Abbiamo detto che è anche la questione economica principale, cioè il nuovo e necessario ambito di intervento finanziario di investimenti di parte pubblica in grado di sollecitare, promuovere e sostenere anche la capacità produttiva più complessiva della società mondiale.

partendo dalla consapevolezza che abbiamo la necessità di salvare il pianeta per salvare noi stessi, perché noi non ci salviamo se non salviamo il pianeta; convinti come siamo che per fare questo, non basta fare azioni di natura formale, anche giuridicamente rilevanti, se non siamo poi coerenti fino in fondo sul piano dei comportamenti; convinti come siamo che questa è una materia che non si può trattare a livello nazionale, che deve essere trattata come fa l'Accordo, che è una grande conquista, che noi ratificheremo con l'impegno che sentiamo rispetto a questo tema.

è anche di ciascuna delle istituzioni, a partire da quelle più piccole che hanno responsabilità di gestione del territorio, di governo delle questioni di natura ecologica: come un Comune gestisce la partita dei rifiuti vale per come noi siamo in grado di rispettare

una responsabilità del singolo cittadino, delle comunità locali, delle comunità regionali e nazionali. Noi chiediamo che da questo punto di vista ci sia una traccia verificabile nella prossima manovra di bilancio. Sono anni che facciamo battaglie sul fronte della sicurezza e manutenzione del territorio e su quello della riqualificazione ambientale, del ripristino e della bonifica di aree compromesse. anni che richiamiamo ad una modalità di gestione anche degli indici di inquinamento nell'attività produttiva industriale, in modo che non siano trattati con provvedimenti di natura giuridica atti a garantire principalmente la produzione industriale piuttosto che la vita. Va cioè capovolto questo questo approccio: prima la vita. Dopodiché adeguiamo i sistemi di produzione industriale e di consumo a quella primaria esigenza di salvezza del nostro ambiente naturale e di noi stessi.

più depresse del Paese, perché hanno le attività industriali più impattanti sotto il profilo della tutela dell'ambiente naturale e dei suoi parametri

per la presenza di pericoli di natura ambientale. Vanno quindi individuate - attraverso studi in tal senso - modalità di produzione coerenti con l'Accordo che stiamo ratificando e che abbiamo già sottoscritto.

viene sottoposto al nostro esame il disegno di legge di ratifica ed esecuzione dell'Accordo di Parigi sul clima, adottato lo scorso dicembre al termine della COP21

L'Accordo entrerà in vigore il prossimo 4 novembre 2016. Altri Stati hanno provveduto alla sua ratifica. Oggi tocca all'Italia e tutti siamo ormai consapevoli di quanto l'attuazione dell'Accordo di Parigi, che sostituirà l'impianto dell'attuale Protocollo di Kyoto, sia essenziale per il raggiungimento degli obiettivi in materia di sviluppo sostenibile. Accordo prevede che le parti dovranno presentare ogni cinque anni i contributi nazionali programmati che intendono progressivamente conseguire. Tali programmi per l'Unione europea prevedono una riduzione delle emissioni di gas ad effetto serra almeno del 40 per cento entro il 2030, obiettivo già fissato dal Consiglio europeo sin dal 2014. Questo limite è stato fissato perché il pianeta si trova in uno *status* di emergenza climatica che rischia di concretizzarsi in un suo surriscaldamento di oltre 4 gradi centigradi, fatto che avrà conseguenze irreversibili per il pianeta stesso e il genere umano e che saranno già visibili fra poco più di mezzo secolo. Tra le possibili ripercussioni potrebbero avverarsi tempeste e inondazioni che si abbatteranno con sempre maggior intensità sulle zone sulle zone costiere del mondo, provocando bibliche migrazioni di milioni di persone, mentre il riscaldamento del clima modificherà le zone forestali e le zone umide del pianeta causando danni, a volte irreversibili, all'intero ecosistema. L'allarme è particolarmente grave nel nostro Paese. Secondo l'analisi dei dati delle temperature, fatta dall'Istituto di scienze dell'atmosfera e del clima del Consiglio nazionale delle ricerche, l'Italia si sta scaldando più velocemente della media globale e di altre terre emerse del pianeta. La tendenza del riscaldamento globale, che si può calcolare valutando non solo i dati di un anno, ma anche l'andamento degli ultimi decenni, è per l'Italia una volta e mezzo quella delle media delle terre emerse e il doppio di quella di tutto il pianeta. Tale dato va ulteriormente studiato e analizzato. Sarà compito perciò del nostro sistema nazionale della ricerca darci utili indicazioni. l'aver approvato ieri il disegno di legge che incentiva gli studi in geologia e in scienze della terra potrebbe contribuire come un primo passo passo verso la strada dell'incentivazione della ricerca e delle analisi dei fenomeni legati alle modificazioni

ridurrebbe significativamente i rischi e gli impatti dovuti al cambiamento climatico. L'Accordo di Parigi doveva essere molto ambizioso e sotto alcuni profili lo è stato. Il fatto che 188 Paesi si siano impegnati, tramite una strategia vincolante, a controllare e limitare le loro emissioni di gas serra indubitabilmente è un risultato storico. Tuttavia, come era già chiaro prima dell'inizio del COP21, non è ancora sufficiente a limitare la crescita della temperatura al di sotto dei 2 gradi centigradi rispetto a quella preindustriale. Per questo motivo il processo di divisione e aggiornamento degli impegni che l'Accordo di Parigi delinea giocherà un ruolo di fondamentale importanza nel promuovere azioni sempre più ambiziose. A questo proposito, il nostro sguardo è già rivolto al prossimo incontro, la cosiddetta COP22, che si terrà a Marrakech dal 7 novembre, durante la quale verranno ulteriormente definiti, in particolare, i modi e i tempi di attuazione dei passaggi intermedi della strategia di Parigi, in modo che questa possa operare operare in maniera efficace. Un aspetto cruciale per il raggiungimento dei traguardi prefissati sarà la mobilitazione delle risorse finanziarie necessarie per permettere ai Paesi in via di sviluppo di definire piani di mitigazione e adattamento,

è stato svolto dal settore privato, che per la prima volta ha assunto impegni rilevanti di riduzione delle emissioni di gas serra, ma anche dalla società civile e dalle istituzioni locali. La complessa problematica investe le responsabilità politiche. Da anni in Italia non si programmano politiche industriali. Oggi scontiamo i ritardi, gli sperperi, l'impreparazione alle nuove sfide che sono eminentemente culturali, vocate al cambiamento e all'innovazione. Oggi l'Italia ha politiche industriali precarie: il controverso caso ILVA in Puglia è emblematico e drammatico al contempo. Il cambiamento non è solo possibile, ma può essere una straordinaria opportunità, mentre la non azione avrà un costo enorme dal punto di vista ambientale (con danni agli ecosistemi), economico (con danni alle infrastrutture e ai processi produttivi) e sociale (con l'aumento del tasso di emigrazione e di mortalità umana dovuta agli effetti dei cambiamenti climatici). Per questo il Governo dovrebbe davvero mettere in pratica una strategia nazionale concreta e incisiva per la riduzione delle emissioni, da un lato, di adattamento ai cambiamenti climatici, dall'altro, mediante l'adozione urgente di provvedimenti diretti a incentivare una maggiore responsabilizzazione dei settori diversi dall'industria, che contribuiscono in misura determinante alle emissioni: i trasporti, l'agricoltura, l'edilizia residenziale, le grandi infrastrutture. In questo contesto, occorrerebbe valorizzare il patrimonio industriale esistente, favorendo, in tutti i settori produttivi e nel terziario, l'adozione di tecnologie che aumentino la compatibilità ambientale dei processi produttivi, l'ecosostenibilità e lo sviluppo di nuove attività produttive in settori più strettamente collegati alla *green economy*.

Signora Presidente, cari colleghi, l'Accordo di Parigi del dicembre 2015, che oggi il nostro Paese è chiamato a ratificare, è finalizzato nei suoi dettagli alla protezione del clima del pianeta.

Riconoscono la necessità di dare una risposta efficace e progressivamente crescente alla minaccia urgente del cambiamento climatico. Riconoscono i bisogni specifici dei Paesi in via di sviluppo, specie specie di quelli particolarmente vulnerabili agli effetti negativi dei cambiamenti climatici. Riconoscono, inoltre, la priorità fondamentale di salvaguardare la sicurezza alimentare e porre fine alla fame. Quest'ultimo punto è stato richiesto a gran voce dalla FAO e raccorda, inoltre, il testo ai primi due grandi obiettivi universali di sviluppo sostenibile. I Paesi firmatari, inoltre, riconoscono che il cambiamento climatico è una questione comune dell'umanità e i Paesi dovrebbero, quando agiscono per affrontarlo, rispettare, promuovere e considerare i diritti umani, il diritto alla salute, i diritti dei popoli indigeni, delle comunità locali, dei migranti, dei bambini, delle persone diversamente abili, di chi è in situazioni vulnerabili e il diritto allo sviluppo, così come l'eguaglianza tra i sessi e l'equità tra le generazioni. I Paesi sottolineano l'importanza di assicurare l'integrità di tutti gli ecosistemi, inclusi gli oceani e la protezione della biodiversità. E sottolineano l'importanza del concetto di «giustizia climatica», quando si agisce rispetto al cambiamento climatico. Tutto questo è contenuto nel preambolo dell'Accordo, che rappresenta anche la base culturale su cui esso si fonda. L'obiettivo prioritario della Convenzione è, quindi, stabilizzare la concentrazione in atmosfera dei gas climalteranti a un livello che eviti una pericolosa interferenza umana nel sistema, salvaguardando l'equilibrio della vita sul nostro pianeta. Certamente l'Accordo per contrastare i cambiamenti climatici incoraggia trasformazioni profonde dei settori industriali, dell'energia, dei trasporti, dell'edilizia, dell'agricoltura, che richiedono in ogni tappa decisioni coraggiose e non facili.

assolutamente procedere ad alcuna riduzione delle emissioni e che toccava ancora ai Paesi sviluppati fare gli sforzi maggiori, allora possiamo dire che l'Accordo di COP21 è davvero storico poiché per la prima volta, riguardo al clima, tutti i Paesi si sono impegnati in maniera attiva per ridurre le emissioni serra. Il testo contiene davvero un obiettivo molto ambizioso, che fino a pochi anni fa sembrava inimmaginabile, e cioè che la crescita della temperatura deve essere bloccata al di sotto dei 2 gradi rispetto all'era preindustriale. Inoltre, i Paesi industrializzati si sono impegnati ad alimentare un fondo annuo da 100 miliardi di dollari (a partire dal 2021, con un meccanismo di crescita programmata) per il trasferimento delle tecnologie pulite nei Paesi non in grado di progredire verso la *green economy*.

Lo stesso presidente Obama, alla vigilia del G20, ebbe a dire che la cooperazione è «la miglior *chance* che abbiamo» e aveva ragione. Se tutti saremo in grado di onorare l'Accordo di Parigi e a rispettare il *target* sulla riduzione delle emissioni responsabili dell'effetto serra, allora avremo fatto fatto un passo verso il vero progresso dell'umanità. È una battaglia che ogni singolo Paese non può fare da solo, anche se si trattasse del più potente e ricco.

Se è vero, com'è vero, che la lotta ai cambiamenti climatici si conduce sul fronte della riduzione delle emissioni in atmosfera, è anche vero che tutto questo passa attraverso un cambiamento radicale nel modo di affrontare il tema dei rifiuti e quello delle emissioni in atmosfera. Infatti, l'affermazione dei principi dell'economia circolare, di cui tanto si parla e sui quali siamo assolutamente d'accordo, volta al recupero della materia, al riciclo, al riuso, costituisce certamente un cambiamento radicale in grado di impattare positivamente sull'ambiente, con meno risorse utilizzate e meno emissioni, sulla filiera di recupero, sulla manifattura, ma anche sui cittadini, con una riduzione di circa il 20 per cento del costo di gestione dei rifiuti urbani (anche questo con un impatto economico rilevante per i cittadini stessi). quanto ci dice la Banca mondiale, le azioni di contrasto ai cambiamenti climatici sono foriere di un aumento del PIL, stimato finora a 1.900 miliardi di euro l'anno,

diciamo che piena e intera esecuzione potremo dare a questo Accordo solo se saremo coerenti e capaci di tracciare una strategia consequenziale sull'ambiente e l'energia, perché solo su questa base potremo essere giudicati credibili sul piano internazionale, ma soprattutto dalle nostre future generazioni.

Il Senato - lo ricordo - il primo dicembre dello scorso anno discusse in questa sede mozioni sui cambiamenti climatici, quando la ventunesima Conferenza del clima di Parigi era già iniziata. Le mozioni erano volte a dare indirizzi al Governo

anche oggi come Paese, perché l'Accordo di Parigi sul clima è stato siglato il 12 dicembre, a conclusione della COP21.

Poi, lo scorso 4 ottobre è stato ratificato dall'Unione europea e da altri sette Paesi membri

Il 4 novembre è qualche giorno precedente l'inizio della COP22 di Marrakech, in Marocco, dove, dal 7 al 18 novembre, si inizierà ancora a discutere di cambiamenti climatici, con particolare riferimento L'Accordo di Parigi ha degli obiettivi che rappresentano una grande sfida che ovviamente tutti devono condividere.

un delta di temperatura all'interno dei 2 gradi rispetto ai livelli preindustriali, con l'impegno, aggiunto positivamente durante la Conferenza di Parigi, di operare attivamente

certamente condivisibile, perché bisogna fermare le catastrofiche conseguenze che da qualche anno si stanno registrando a causa del riscaldamento globale e della temperatura media del

estesi e talvolta irreversibili per le popolazioni e gli ecosistemi. L'obiettivo del contenimento dell'aumento della temperatura entro i 2 gradi (possibilmente entro 1,5 gradi) non può che passare attraverso questo Accordo di carattere universale, globale e durevole, che deve avere degli obiettivi scadenzati nel lungo termine: un Accordo che deve essere assolutamente trasparente e tutti

avranno il testo, come ha giustamente denunciato all'inizio della seduta il collega Azzollini - sarà presente, scritto nero su bianco, il piano di investimenti di 4 miliardi di euro da qui al 2020 che, durante la Conferenza di Parigi, davanti a una vetrina mondiale,

che ogni Paese adotta per la produzione di energia: c'è chi la produce ricorrendo esclusivamente alle fonti fossili (in particolare, il carbone); ci sono poi altri Paesi, come il nostro, che ricorrono invece all'utilizzo di fonti rinnovabili

Approfitto della presenza del ministro Galletti, per ricordare (a nome del Gruppo della Lega Nord) che il Governo italiano, posto che dovrà ovviamente monitorare e operare fattivamente

infatti, «l'Italia è il Paese dell'Unione europea che segna il *record* del numero di morti prematuri rispetto alla normale aspettativa di vita per l'inquinamento dell'aria».

sono gli agenti chimici *killer* sotto accusa, per questo tristissimo primato: le micropolveri sottili, il biossido di azoto e l'ozono.

Stiamo parlando - guarda caso - delle aree del Paese maggiormente antropizzate, dove incide maggiormente il riscaldamento domestico, a cui si ricorre per le fredde temperature invernali, ma dove c'è anche il maggior congestionamento del traffico automobilistico, anche e soprattutto a causa dell'insufficienza delle infrastrutture stradali. Concludo dicendo che va bene, dunque, la tutela dell'ecosistema

che presenta delle criticità pesanti in Pianura Padana, occupandoci anche della tutela della salute umana degli abitanti di quella parte importante del Paese. *(Applausi del senatore

provvedimento "destinazione Italia", meglio detto lo "spalma incentivo"; come se non fosse il Parlamento che ha votato lo "sblocca Italia" delle trivelle e degli inceneritori; come se fossimo in un altro Paese e ci fossimo resi conto di quale sia il problema; come se non fossimo

La Commissione europea, nella relazione che accompagna la proposta di modifica del regolamento n. 525 che abbiamo avuto in esame in Commissione fino all'altro giorno, sottolinea come, con le attuali tendenze, le emissioni di gas serra non potranno diminuire sufficientemente per centrare l'obiettivo di una riduzione annuale del 30 per cento rispetto al 2005 e quindi non verranno centrati gli obiettivi di Questo è un fatto, è un dato, è una dichiarazione. scritto, nero su bianco, che non stiamo andando nella giusta direzione e oggi, con grande ritardo, andiamo a ratificare l'Accordo. Giusto, ben venga, ma dobbiamo essere coscienti del ritardo, coscienti del fatto che non stiamo andando nella giusta direzione.

Eppure, noi riusciamo a dirci soddisfatti se nel 2014 e 2015, per la prima volta da molti anni, la crescita delle emissioni a livello mondiale - badiamo anche in presenza di una crescita a livello globale. Questo, però, è un dato che viene registrato soltanto osservando i dati positivi dei Paesi in via di sviluppo,

È questa la situazione in cui ci troviamo. Siamo passati dal 1990 ad oggi da 38 gigatonnellate di CO2 equivalente a 54 gigatonnellate di CO2 equivalente. Questo è il *trend*, questo è il nostro cammino.

Abbiamo raggiunto a livello mondiale 286 miliardi di dollari di investimento, ma è stato solo grazie ai Paesi in via di sviluppo che hanno superato di gran lunga i cosiddetti Paesi industrializzati.

hanno registrato un dato veramente allarmante di un decremento crescente negli investimenti, che nel 2015 ci riporta ai livelli del 2008. Questo siamo noi. Nel 2013 l'Europa ha perso definitivamente la *leadership* mondiale di investimenti nelle tecnologie *green*

L'Unione non è attualmente sulla strada per poter conseguire il *target* del pacchetto 2030. Inoltre, i *target* in rinnovabili e di efficienza del pacchetto del pacchetto 2030 non sono sufficienti a conseguire il *target* di meno 40 per cento di gas serra che si è data Parigi. Questa fonte proviene dalla Fondazione di sviluppo sostenibile. E quel meno 40 non è valutato neanche sufficiente perché, per raggiungere gli obiettivi di Parigi, ossia contenere il surriscaldamento a un grado e mezzo, sembra

Si registra, invece, un incremento di CO2 in controtendenza con gli altri anni. E le proiezioni al 2020 e al 2030 prevedono ulteriori preoccupanti incrementi. Noi tenderemo, cioè, verso il 2020 e il 2030 ad aumentare le emissioni di CO2 e non a diminuirle. Questo è il *trend*.

si invitano gli Stati membri a rivedere al rialzo i propri impegni di decarbonizzazione, per rispondere alla sfida di Parigi. È anche il Parlamento europeo, quindi, che riconosce che non stiamo andando nella giusta direzione. La nuova *road map*, secondo la Fondazione, dovrebbe prevedere per l'Europa nel 2030 una riduzione del 50-55 per cento di emissioni rispetto al 1990, contro il 40 per cento che ci eravamo prefissato. Quindi, dobbiamo assolutamente accelerare le azioni. In Italia, è necessario attivare

è dovuto anche alle scellerate scelte legislative che hanno causato grande danno alle fonti energetiche rinnovabili e grande favore al vecchio fossile.

i risultati delle azioni si calcolano. Ci sono delle tabelle, ci sono delle statistiche, ci sono degli studi che ci parlano e con chiarezza ci mostrano il risultato delle nostre azioni.

andando così meglio della media europea di Spagna, Francia e anche Germania. Poi però le rinnovabili hanno avuto cali

a soli 122 ktep aggiuntivi del 2015. Il rapporto dei numeri parla chiaro: non sono chiacchiere, non è sofismo e non è retorica. I numeri ci dicono dove stiamo andando. occorre una nuova SEN 2030, con *target* capaci di avvicinarci all'impegno di Parigi: Parigi: ridurre le emissioni, ridurre i consumi finali e aumentare il consumo finale lordo di rinnovabili elettriche. Secondo l'IPCC, il *carbon budget* residuo al 2100, nello scenario a 2 gradi, è pari a non più di 1.100 Gt; a oggi sono state emesse oltre 2.000 Gt. Secondo l'IEA per rispettare il *carbon budget* a 2 gradi, un terzo delle riserve di petrolio, metà delle riserve di gas e l'80 per cento delle riserve di carbone dovrebbero rimanere interrate. il *carbon budget*, rivisto nello scenario a 1,5 gradi, è circa la metà di quello a 2 gradi,

Ci appare quindi opportuna questa ratifica, anche se tardiva, ma ci sembra già urgente un progetto di revisione dei *target* europei e nazionali delle emissioni di gas a effetto serra. Noi dobbiamo davvero (e doverosamente)

siamo gli ultimi, ma non possiamo certo vantarci al riguardo. L'Accordo di Parigi fissa nuovi e più sfidanti obiettivi per i Paesi firmatari, fra i quali l'Unione europea contenere l'aumento della temperatura media globale ben al di sotto dei 2 gradi rispetto ai livelli pre-industriali, perseguendo tutti gli sforzi necessari per limitare tale aumento a 1,5 Questo nuovo obiettivo è molto più impegnativo di quanto si potrebbe credere: fermare l'innalzamento della temperatura globale a 1,5 gradi in luogo di 2 significa all'incirca dimezzare i quantitativi di gas serra che potranno essere complessivamente emessi in atmosfera nel resto del XXI secolo. Per rispettare l'Accordo di Parigi, l'Unione europea - e quindi l'Italia - dovrà rivedere in modo significativo i propri impegni climatici al 2030. Questi nuovi obiettivi da soli, tuttavia, non bastano. Sarà necessario mettere in campo efficaci politiche e misure per la loro attuazione che non potranno essere la semplice prosecuzione di quanto già in essere. non potranno essere la semplice prosecuzione di quanto già in essere. L'elevato grado di ambizione concordato a Parigi richiederà infatti approcci e strumenti innovativi in grado di imprimere l'accelerazione necessaria per realizzare un svolta sostenibile ai fini dell'implementazione di quanto Il nostro Paese, per essere in grado di cogliere l'enorme potenziale della transizione in corso e la grande opportunità di rilancio economico ed occupazionale che rappresenta, ha necessità di definire un quadro certo di medio e lungo periodo, con scelte chiare in grado di tracciare i lineamenti di un nuovo programma nazionale, capace di indirizzare gli investimenti, non solo del settore energetico ma di tutti i comparti coinvolti nella transizione. Lo scenario alternativo vedrà altrimenti la perdita di competitività delle nostre imprese nel mercato globale del futuro, dove le soluzioni e le tecnologie *green* giocheranno un ruolo preponderante nei diversi settori; energetico, edile, trasporti, pianificazione urbana, servizi, agricoltura, silvicoltura ed altri usi del suolo. Sarebbe utilissimo offrire fondamento giuridico all'attuazione dell'articolo 6 dell'Accordo, che riguarda la collaborazione internazionale (su tutti i temi, incluso mitigazione ed adattamento) e che prevede sia meccanismi di mercato che non di mercato (leggi, obblighi, divieti). Questo quadro, per realizzarsi, dovrà essere economicamente sostenibile. Da questo punto di vista, i classici meccanismi di incentivazione a singhiozzo hanno mostrato spesso una mancanza di efficienza e di efficacia. Essenziale quindi risulta essere una riforma di sistema che garantisca la finanziabilità di tale transizione sostenibile. L'articolo 4 del disegno di legge di Gli eventuali oneri finanziari conseguenti ai contributi determinati a livello nazionale, previsti dall'articolo 4, paragrafi 2 e 3, dell'Accordo di cui all'articolo 1, saranno autorizzati con appositi

di questi processi, ma l'Italia sta perdendo il treno della messa in visibilità internazionale e del suo straordinario patrimonio di *green economy*, *soft economy* e competenze industriali e territoriali. In base alle conclusioni del Consiglio europeo, l'obiettivo dovrà essere raggiunto collettivamente dall'Unione nel modo più efficace possibile, in termini di *cost*, mediante riduzioni delle emissioni sia nei settori che rientrano nel sistema di scambio di quote di emissioni ETS, sia negli altri settori, rispettivamente pari al 43 e al 30 per cento rispetto al 2005; e qui vi è poi la frase cruciale, la frase che secondo me ci insulta:

Stato si autosostiene con la *green economy* e ha un alto PIL, come è possibile ragionare in questo modo? Possiamo almeno fare il bene di tutti e ragionare in un modo virtuoso, senza avvantaggiare *semper chi tai*, come si dice a casa mia? Non è il PIL totale, ma è il PIL prodotto e ottenuto, decurtato della parte ottenuta con la *green economy* del PIL prodotto in modo autosostenuto. È qui infatti il problema. Va bene che ci siano proporzionalità in base al PIL, ma non il PIL totale. totale. Noi, qui, Ministro, dobbiamo alzare la voce, dobbiamo farci sentire. Qui ci si concentra solo sugli oneri finanziari e non sui processi concertativi per l'attuazione, già previsti a Kyoto. Qui noi ci muoviamo dopo gli altri, ponendoci solo questo tema oneroso e non quello dei vantaggi, consegnando uno strumento tipicamente e marcatamente nazionale consegnando uno strumento tipicamente e marcatamente nazionale come il contributo determinato a livello nazionale a un opaco negoziato europeo, che ha partorito un impegno solo numerico, senza alcun elemento di attuazione, e che non intercetta in alcun modo evidente il posizionamento competitivo e i fabbisogni dell'Italia. Un primo passo miliare dovrebbe essere una revisione della fiscalità in chiave ecologica che, nel rispetto della neutralità fiscale, modifichi in modo profondo le convenienze degli investimenti verso tecnologie e interventi a bassa emissione di carbonio. Diversi sono gli strumenti e le strategie che possono essere messi in atto, come il *carbon pricing* o interventi di riallocazione ed eliminazione dei sussidi dannosi, fino a facilitazioni di accesso al credito e strumenti di sostegno economico tarati sulle singole tecnologie. Certo, queste sono visioni lungimiranti della gestione di un'economia, ma è solamente con una visione lungimirante che si possono coniugare salvaguardia dell'ambiente, convenienza di mercato, innovazione tecnologica e sviluppo per il nostro Paese. porti avanti il suo genio e la sua ricerca perché ne ha una concentrazione unica al mondo, ma serve una consapevolezza che forse qui non abbiamo. Serve il coraggio di alzare la testa con dignità davanti all'Europa;

qualche ragionamento aulico e anche ridondante; viceversa abbiamo ascoltato degli interventi assolutamente catastrofisti, che a mio avviso non si confanno al merito del provvedimento, ma soprattutto non rendono atto di quello che ha fatto il nostro Governo e soprattutto lei che in questi anni nelle trattative internazionali con gli altri Paesi dell'Unione europea (tra l'altro sono testimone di trattative anche con Paesi non facenti parte dell'Unione europea) ha sempre avuto un ruolo da protagonista, soprattutto di chi guarda al futuro con intelligenza e lungimiranza. Abbiamo sentito parlare di scomparsa della biodiversità, di distruzione della fauna globale (a proposito di fauna globale, sappiamo come lo *stock* delle risorse ittiche sia in rapida caduta non solo nel Mediterraneo, ma anche negli oceani), di diminuzione di tutte le risorse sistemiche che permettono la vita di tutte le specie e anche dell'uomo. A dire la verità, c'è un tema che a me sta molto a cuore in materia di cambiamenti climatici ed è relativo alle dirette conseguenze che tra l'altro subiamo noi italiani nel Mediterraneo, in particolare noi siciliani, che è quello dell'enorme numero dei migranti ambientali e climatici. Dico questo proprio qui in quest'Aula, sperando di cogliere l'attenzione dei colleghi - che peraltro rispetto - della Lega Nord e di altri partiti che sul tema della immigrazione a mio avviso talvolta sono un po' distratti o addirittura un po' faciloni. Il tema dei migranti climatici è fondamentale: ci sono più migranti climatici che migranti da guerra o da altri fenomeni. Quanto sta accadendo nel Centro Africa o nell'Africa subsahariana

Le popolazioni del Nord, quando c'erano le piccole glaciazioni, scappavano verso i Paesi mediterranei: questo dà ragione delle invasioni barbariche. I popoli dei Paesi scandinavi scapparono in quel periodo

nei confronti del quale noi popolazioni europee abbiamo un debito: il debito dello sfruttamento che per secoli ha garantito alle popolazioni occidentali e dopo del Nord America un tenore di vita e di crescita che sicuramente è stato compiuto utilizzando le risorse e le materie prime di altri Paesi che non solo sono stati deprivati di quelle risorse e materie prime, ma che oggi ne stanno subendo le conseguenze. Ed è proprio per questo motivo che noi plaudiamo all'iniziativa del Governo: perché, al di là della ratifica di oggi, che rende atto dello stanziamento del Fondo verde per il clima, la ratifica che andiamo ad approvare in perfetta continuità con quanto fatto a Durban, a Doha e a Parigi, con l'accordo di Marrakech entrerà nel vivo ed entrerà assolutamente nella direzione di un accordo globale di tutti i Paesi. L'obiettivo è quello di un accordo solidale che riesca a controbilanciare l'interesse dei Paesi forti più industrializzati con i Paesi deboli, e che riuscirà in un certo qual modo anche ad abolire quel differenziale di convenienza che si è creato in altri Paesi che nel passato non avevano aderito a questi accordi internazionali e che di fatto ha penalizzato le economie dei Paesi occidentali e anche le economie dei Paesi trasformatori come il nostro. nostro. Signor Ministro, non voglio assolutamente dilungarmi, perché ancora altri dopo di me interverranno e seguiranno anche le dichiarazioni di voto. Sicuramente bene ha fatto il nostro Governo: l'Italia è stata protagonista in Europa, e chi era a Parigi ha toccato

mondiale, l'agenzia meteo dell'ONU, ha annunciato che le concentrazioni di anidride carbonica del pianeta nel 2015 hanno stabilmente superato la soglia (psicologica) delle 400 parti per milione. Le concentrazioni di CO2 che osserviamo oggi sono le più alte da circa un milione di anni, come finora riscontrate dagli studi paleoclimatici. Questo cambiamento nella composizione dell'atmosfera, assieme ad altri stravolgimenti dei cicli biogeochimici naturali, ha portato a definire la presente epoca come Antropocene (la definizione si deve al Paul Crutzen, Nobel della chimica), e cioè una nuova era geologica in cui le attività dell'uomo sono diventate determinanti per il clima mettendo fine all'Olocene, era nella quale si è sviluppata la nostra specie. Ricordo che la CO2 è il più importante dei gas ad effetto serra, ma non è l'unico. Vanno aggiunti altri gas che, pur in concentrazioni inferiori, danno un contributo ulteriore al riscaldamento globale (come il metano, il protossido d'azoto, i gas fluorurati, e altri ancora), mentre va sottratto il contributo di raffreddamento degli aerosol (particolato fine) che hanno invece un effetto opposto, riflettendo la luce del sole, quindi raffreddando il pianeta. Questi contributi possono essere espressi in termini di CO2 equivalente e, da questo punto di vista, le concentrazioni dei gas a effetto serra sono in realtà prossime ai 450 ppm, ma con l'effetto di raffreddamento degli aerosol scendiamo a circa 410 ppm equivalenti. Ricordiamo che a 430 ppm la probabilità di superare gli 1,5 gradi è già superiore al 50 per cento, mentre la soglia dei 2 gradi viene superata con 530 ppm. Ci rimane quindi poco tempo per agire seriamente: le emissioni di gas serra devono scendere molto rapidamente. Ciò che finora ha spinto maggiormente questa dinamica negativa dalla rivoluzione industriale ad oggi è - ricordiamolo ancora una volta - l'impiego dei combustibili fossili, che hanno alterato pesantemente la dinamica del ciclo naturale del carbonio, rimettendo in circolo grandi quantità finora rimaste sottoterra in forma di carbone, petrolio e gas naturale. Le emissioni complessive dal settore della produzione di energia e cemento superano i 35 miliardi di tonnellate di CO2 all'anno. Il motivo per cui le concentrazioni vanno aumentando è anche dovuto al fatto che la capacità di assorbimento della biosfera - foreste e oceani - non arriva alla metà di quello che viene emesso, e, siccome la CO2 permane mediamente in atmosfera per tempi superiori al secolo, questa va accumulandosi producendo un aumento delle temperature. Peraltro, l'assorbimento di CO2 da parte degli oceani - il gas viene fissato dalle alghe - sta contribuendo ad acidificare i mari, fenomeno che desta fortissime preoccupazioni tra gli esperti per le inevitabili conseguenze sull'ecosistema marino mondiale. Per evitare il peggio - scenari di aumento della temperatura superiori ai due gradi centigradi - è necessaria una rapida inversione di tendenza. L'Accordo di Parigi, raggiunto dopo venticinque anni di confronti sterili, ha sì fissato un quadro politico generale, ma gli impegni volontari presi finora non sono ancora sufficienti. La quantità di emissioni di CO2 che ci porterebbe oltre la soglia dei due gradi centigradi è stata stimata in 1.000 miliardi di tonnellate e a tutto il 2011 già metà di questa quantità era stata emessa; per questa ragione le emissioni andranno pressoché azzerate nella seconda metà del secolo. Vedremo se la COP22 manterrà la dinamica dell'Accordo di Parigi che sarà appena entrato in vigore (tra l'altro con un tempo quasi *record* e mai visto negli accordi ambientali internazionali) e cioè se farà progressi la revisione degli impegni volontari che deve procedere più rapidamente. Per evitare il peggio non mancano né la tecnologia, né le risorse finanziarie: quello che scarseggia è il tempo e soprattutto la volontà politica. Mi rivolgo al Governo, nella persona del ministro Galletti, che noi riteniamo troppo assente su questi argomenti: la natura non sente ragioni politiche. Servono risposte che rimuovano le cause. Serve una visione che il Governo non ha, diversa del futuro, degli strumenti di produzione e dei beni di consumo che non impieghino più energie fossili e cemento ma risorse naturali e sostenibili. cari cittadini - che se la effettuassimo genererebbe centinaia di migliaia di nuovi posti di lavoro. Lo voglio sottolineare: la conversione industriale non serve solo a salvare il pianeta, ma genererebbe anche centinaia di migliaia di nuovi posti di lavoro, di nuovi posti di lavoro, ridando dignità a milioni di persone che oggi vivono in condizioni di povertà e di incertezza. Ma, a oggi, la politica del Governo italiano non sta rispondendo adeguatamente Per essere ancora più chiari, Governo e cittadini, stiamo continuando a perdere i treni del presente e del futuro. Ci siamo già dolorosissimamente persi il treno del fotovoltaico, tecnologia nella quale eravamo tra i *leader* all'inizio, e ora rischiamo di perdere il treno delle auto elettriche: uno *tsunami* in arrivo, come lo definiscono addirittura le agenzie di *rating*, e noi non e noi non ci stiamo preparando. Gli altri Paesi si stanno preparando, sono più attivi di noi; noi continuiamo ad avere una visione molto miope, siamo gli ultimi della classe dei 28 Paesi europei per quanto riguarda l'incentivazione delle auto elettriche. Stiamo perdendo anche questo treno, Ministro. Siamo ugualmente fermi di fronte alla necessaria conversione dalla petrolchimica alla chimica verde (lacche, colle, vernici, gomme, resine, plastiche e chi più ne ha più ne metta; anche fertilizzanti e antiparassitari). Lasciamo che siano solo pochi soggetti privati a fare da apripista, ma ancora una volta con una politica italiana assente.

Ricordo che un'importantissima norma per liberalizzare i consorzi di riciclaggio è ferma all'interno del disegno di legge concorrenza, fermo ancora una volta non per colpa della Costituzione, ma con la scusa della Costituzione, mentre la colpa è ovviamente della maggioranza che fa orecchie da mercante e non calendarizza La vostra politica, la politica della maggioranza è ferma anche sulle misure per riutilizzare la filiera agricola (legno e boschi), e boschi), che può portare altri 450.000 posti di lavoro (dati degli organismi di settore). Sono misure che servono sia per la parte ambientale di cattura della CO2 e di stabilizzazione del suolo sia per gli utilizzi industriali

Per farlo dobbiamo proporre loro anche soluzioni per quanto riguarda il problema dell'incapienza e del mero finanziamento. Infatti, se non ci sono capienza fiscale e disponibilità economica ovviamente questo risultato non verrà raggiunto. Solo facendo buone politiche subito sui suddetti comparti che ho brevemente richiamato rispetteremo veramente gli impegni sottoscritti prendendo i classici due piccioni con una fava: salvaguarderemo l'ambiente e creeremo centinaia di migliaia di posti di lavoro. Ministro, dobbiamo però agire subito. Siamo già in fortissimo ritardo rispetto agli altri Paesi.

Signor Presidente, onorevoli colleghi, rivolgo un saluto cordiale al ministro Galletti, che ci ha rappresentato alla COP21 di Parigi e, come diceva il collega Marinello, lo ha fatto dimostrando che l'Italia non vuole essere un Paese

lo possiamo dire in relazione al fatto che avremmo voluto che la rappresentanza politica mondiale recuperasse le iniziative europee ben prima di quanto ha fatto nell'ambito della ratifica sottoscritta proprio dai due Paesi che inizialmente

di partire insieme con le politiche di efficientamento e di riduzione delle emissioni in atmosfera possiamo tranquillamente dire che siamo stati in ritardo come Paesi europei soprattutto rispetto al

L'Europa è stata - voglio dirlo - un esempio positivo, un elemento di sfida sul tema delle emissioni in atmosfera. Ciò ha permesso agli Stati Uniti d'America, con Obama, di partire, già dal 2009 con la COP15 di Copenaghen, accelerando sull'importanza di condividere questa nuova linea strategica funzionale alla salvaguardia del pianeta, ma anche alla qualità del benessere dei cittadini che in questo pianeta abitano, nella riduzione delle emissioni in atmosfera.

un dato che credo debba essere consegnato perché di particolare rilievo: abbiamo 14,3 tonnellate di petrolio equivalente per ogni milione di euro prodotto; siamo, dunque, ben al di sotto di Spagna, Germania e Francia, con 312 tonnellate per milioni di euro prodotto. Siamo sotto qualunque altro Paese europeo,

in tecnologie pulite abbondantemente superiore a tutti gli altri Paesi europei. Concludo con le 107 tonnellate di anidride carbonica, la famigerata CO2 equivalente per milione di euro prodotto. Anche in questo caso siamo primi in Europa con 50 tonnellate in meno della Germania, escludendo la Francia che, com'è noto, con il nucleare parte da un vantaggio competitivo limitato alle emissioni in atmosfera. Siamo stati un esempio positivo ma non ce ne vantiamo; lo diciamo perché abbiamo ascoltato una serie di pessimismi che superano abbondantemente i pessimismi della ragione. PRESIDENTE.

dell'ONU, la più grande convenzione per la riduzione di temperatura mai raggiunta a seguito dell'uso degli idrofluorocarburi per il funzionamento di frigoriferi e impianti di condizionamento. Solo questo prevedrà una riduzione, dal 2017 in avanti, di mezzo

come tutti i Paesi traino, dobbiamo essere un esempio positivo per forzare la mano, per spingere l'acceleratore, per fare in modo che il pacchetto clima-energia come il pacchetto sull'economia circolare raggiungano i loro scopi in tempi rapidi, producendo gli effetti auspicati da tutti noi. Rivolgo un ringraziamento particolare a chi, in questi anni, ha voluto che l'Italia rappresentasse il meglio per quanto riguarda il tema delle energie rinnovabili e della riduzione delle emissioni in atmosfera.

anche io, a nome del Governo, la solidarietà e la vicinanza ai Comuni e ai cittadini colpiti questa notte dal terremoto, riproponendo l'intenzione del Governo di continuare nell'azione di emergenza e di ricostruzione nelle zone

rispetto dell'economia dei lavori, mi esenta dallo svolgere la replica. Rimango chiaramente a disposizione di tutte le Commissioni qualora ritengano di dover approfondire gli argomenti riguardanti l'Accordo di Parigi.

C'è bisogno di finanziare gli interventi di decarbonizzazione? Ci sono circa 14 miliardi di euro che ogni anno le nostre tasche tirano fuori per il carbone, per il petrolio e per tutte queste cose.

vi siano tutti i presupposti perché si faccia presto ma anche impegnando il Governo a mettere in atto politiche industriali che tengano conto, ovviamente, della necessità di una forte riduzione dei gas serra, il tutto il tutto vocato ad una inclinazione nazionale a favorire la *green economy*.

Si deve poi rilevare la difficoltà di siglare questo tipo di accordi con Paesi che sulla carta sono in via di sviluppo, ma che a tutti gli effetti sono delle vere e proprie potenze mondiali

Certo, tutto è perfettibile e migliorabile, ma non possiamo sottacere che l'Accordo prevede, per la prima volta, che i Paesi dovranno fare un vero e proprio inventario delle loro principali fonti di inquinamento e condividerle con il resto del mondo. Dovranno monitorare le emissioni di carbonio, con metodi di misura *standard*, e riferire periodicamente sui progressi in atto per ridurre tali emissioni. L'Accordo prevede anche un Fondo di investimento pubblico e privato per un totale di almeno 100 miliardi di dollari l'anno, per aiutare i Paesi a basso reddito a proteggersi dalle minacce legate al cambiamento climatico globale e ad investire nelle energie pulite in modo da migliorare la vita dei loro abitanti. Credo, in conclusione, che i lati positivi di questo Accordo superino di gran lunga i tratti negativi o deficitari.

Presidente, signor Ministro, colleghi, anzitutto comunico il voto favorevole del Gruppo per le Autonomie-PSI-MAIE al disegno di legge n. 2568 di ratifica dell'Accordo di Parigi sui cambiamenti climatici, firmato lo scorso 12 dicembre Si tratta di un Accordo che è sicuramente storico per almeno due ragioni: gli obiettivi che si pone, ovvero contenere in due gradi centigradi l'aumento della temperatura del pianeta (con la possibilità, anzi l'auspicio di contenerlo in 1,5 gradi) e la quantità dei Paesi che lo hanno sottoscritto e già ratificato. Per raggiungere questo obiettivo vi è stato un proficuo lavoro di coordinamento, negoziato e infine accordo, che ha visto come protagonista l'Unione europea e questo fa piacere in questo momento di crescente euroscetticismo.

ad una rapida ratifica e per questo motivo siamo qui: proprio per questa rapida ratifica. I prossimi anni saranno decisivi per raggiungere gli obiettivi prefissati e già l'appuntamento di novembre a Marrakech è un primo importante momento di verifica dei risultati conseguiti. Questo accordo è comunque solo il primo passo di un lungo percorso che tutti insieme, tutto il mondo, dovranno necessariamente compiere nei prossimi anni.

che, appunto, ci ha fatto correre il rischio di partecipare a Marrakech solo come osservatori. E perché si è tentato di rallentare fino all'ultimo il percorso di ratifica?

l'idea di voler tutelare la propria strategia di sviluppo basata sul carbone, noi mascherandoci dietro il principio un po' ambiguo dell'equità, abbiamo tentato dietro le quinte di abbassare l'asticella dei nostri impegni

per la riconversione ecologica del nostro Paese mettendo in atto politiche davvero di riduzione delle emissioni, che rischia di penalizzare il nostro Paese. Dovremmo invece essere in prima linea

costellati da dichiarazioni colme di intenti da un lato e provvedimenti gravissimi dall'altro. Vorrei ricordare qui alcune scelte che sono state fatte e che sono in controtendenza rispetto all'accordo e agli impegni che ci dobbiamo assumere con questa ratifica.

la Conferenza di Parigi ha prodotto un Accordo che riteniamo caratterizzato da molti limiti e anche molte timidezze, ma che, tuttavia, ha riunito la comunità internazionale sotto l'impegno vincolante di contenere il riscaldamento globale sotto la soglia dei 2 gradi rispetto ai livelli preindustriali, perseguendo gli sforzi per limitare tale incremento a 1,5 gradi. Le contraddizioni esistono nell'Accordo: i singoli punti del testo non risultano vincolanti e l'impianto risente della comune tendenza a limitarsi allo strumento dei contributi volontari.

direttamente al nostro Governo perché si metta in campo davvero una progettualità diversa, senza ambiguità. Occorre, per essere chiari, formulare con nettezza l'obiettivo di escludere escludere progressivamente le fonti fossili dal modello di sviluppo, raggiungendo la neutralità emissiva nel 2050. Occorre, ministro Galletti, chiarezza una volta per tutte: occorrono impegni seri sulla fiscalità ambientale per ridurre ed eliminare tutti i sussidi alle fonti fossili e occorre una strategia energetica nazionale in linea, non in contraddizione, con i percorsi di decarbonizzazione. Occorrono a questo punto impegni seri e veri, non le solite ambiguità di cui, appunto, vi state rendendo responsabili. Questo Governo, purtroppo, si ricorda spesso delle questioni ambientali quando sono utili

ma penso che servano e serviranno una discussione vera e impegni precisi da parte del Governo, che, purtroppo, finora ha dimostrato un'impostazione sulle politiche ambientali forse degna della prima rivoluzione industriale. *(Applausi

e a mio avviso è un ottimo risultato raggiunto. Non ci accontentiamo, caro Ministro, e buttiamo il cuore oltre l'ostacolo. Personalmente ho sentito musica per le mie orecchie, quando si è parlato di decarbonizzazione perché, essendo un grande fautore della civiltà rurale, un po' da conservatore (se non addirittura da reazionario), che il modello di sviluppo fosse quello e che gli errori in questo Paese siano stati tantissimi, a cominciare dalla riforma agraria. Nulla di più sostenibile del grande feudo meridionale dal punto di vista ambientale e in questo posso in parte

Presidente, colleghi, signor Ministro, voteremo favorevolmente alla ratifica di questo Accordo. Come già detto dai miei colleghi, lo faremo con alcuni «ma» e con alcune grandi perplessità. Se è vero che la lotta ai cambiamenti climatici costituisce uno degli obiettivi dell'Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile, entrata in vigore il primo gennaio del 2016, mi chiedo: chi stabilisce questi obiettivi? Chi è che stabilisce le tempistiche? E con quale partecipazione nei processi decisionali? Ebbene, credo che nel XXI secolo sia autentico e realistico programmare gli obiettivi e il percorso dello sviluppo sostenibile - se così lo vogliamo continuare a chiamare per comodità solo attraverso processi decisionali partecipati e attuati con forme di democrazia diretta. La democrazia delegata su questi temi - e anche su altri, a dire il vero - ha fatto il suo tempo. Mi chiedo: quale credete voi sia stato il primo grande processo di sviluppo sostenibile nella storia dell'umanità? Credo di poter dire che sia stata la scoperta del fuoco. La scoperta del fuoco e la capacità di poterlo replicare autonomamente hanno rappresentato il primo vero rapporto tra uomo ed energia. La gestione sostenibile di quella forma di energia primitiva ci ha evitato una prospettiva sociale poco gradevole e naturalmente non parlo solo dei cibi crudi che ancora oggi ci troveremmo a mangiare senza la scoperta del fuoco. In più, il dominio dei nostri antenati sul fuoco, la produzione diretta e, soprattutto, la distribuzione partecipata e liberalizzata di quella energia dei primordi hanno prodotto la partenza, lo *start* della crescita collettiva. E allora, chi gestisce l'energia ha un grande potere, perché l'energia è il motore principale di ogni forma di sviluppo economico e sociale. Se questo potere però non lo tengo per me, ma lo ridistribuisco equamente nella società nella quale vivo, ecco che ho creato nei fatti le condizioni per uno sviluppo economico sostenibile. Se poi questa stessa energia è prodotta con elementi naturali - un fulmine che incendia un albero, due acciarini che si sfregano, il sole che illumina un pannello fotovoltaico, il vento che muove un'elica - lo sviluppo diventa doppiamente sostenibile. In primo luogo, perché riduciamo lo sfruttamento di fonti energetiche con alto impatto sull'ambiente; luogo, perché consentiamo l'autoproduzione e distribuzione di energia da fonti rinnovabili e naturali da parte di singoli cittadini, famiglie e aziende. e aziende. Provate ad immaginare per un attimo cosa sarebbe successo se l'accensione del fuoco in epoca primordiale non fosse stata frutto di un processo naturale e di semplice accesso, ma di una tecnologia complessa in mano ad un piccolo gruppo cavernicolo di potere, così come è oggi lo sfruttamento delle fonti fossili in mano a poche, grandi multinazionali. Ebbene, credo che avremmo avuto una società primordiale che, anziché crescere in maniera sostenibile e diffusamente sul pianeta, avrebbe anticipato di migliaia di anni la nascita della società capitalistica. società nella quale un gruppo di potere, gestore verticistico dell'energia necessaria a muovere il mondo, condiziona i Governi e le economie del mondo stesso. Mi rendo conto che la rivoluzione industriale, resa possibile dall'uso delle fonti fossili, ha permesso di raggiungere un livello di tecnologia elevatissimo, consentendo all'uomo un salto di conoscenza impressionante. Mi rendo anche conto che una parte del mondo grazie a petrolio e gas ha raggiunto livelli economici, sociali e culturali impensabili appena un secolo fa. Anche grazie alle risorse derivanti dallo sfruttamento di fonti fossili in alcune aree del pianeta è finito il colonialismo economico e culturale imposto per secoli dall'Occidente. Per questi Paesi però, riuscire a replicare un modello economico e culturale subito per secoli non significa percorrere la strada giusta per il bene del proprio popolo. E allora oggi, sulla terra e nel ventunesimo secolo, non è più pensabile che una oligarchia economica e politica decida delle sorti del pianeta *(Applausi dal Gruppo M5S)*, senza considerare le tensioni sociali nelle mille e mille *banlieue* del pianeta stesso, senza considerare le guerre combattute in nome del petrolio e i milioni di migranti che un modello economico basato sul profitto per il profitto sradica dalla loro terra e proietta verso terre sconosciute. Questi sono i nuovi schiavi di un modello economico che non sta facendo i conti con l'immediato futuro, un futuro nel quale la semplificazione della tecnologia occorrente per fare economia e produrre energia inevitabilmente renderà renderà sempre più universali, diffusi, partecipati e sostenibili i modelli decisionali e le scelte conseguenti. io credo fermamente che nel terzo millennio le scelte per un adeguato e autentico sviluppo sostenibile del pianeta e dei popoli che lo abitano non possano più essere imposte dall'alto o da forme di democrazia delegata. Sono convinto che lo sviluppo sostenibile possa essere guidato efficacemente soltanto da forme di democrazia diretta. Mi rendo conto che non è facile trovare formule che spostino il governo dei Paesi da una democrazia delegata a una democrazia diretta. Non vedo però altra strada: lo sviluppo sostenibile del pianeta ha bisogno di autoproduzione e distribuzione dell'energia e di decisioni derivanti da forme di democrazia diretta. alla conclusione, ritengo doveroso sottolineare che la democrazia diretta è inevitabile. Questo è quanto il Movimento 5 Stelle sta proponendo al Paese dall'inizio di questa legislatura ed è uno dei cambiamenti politici necessari e non più rinviabili,

sul contrasto ai cambiamenti climatici, anche se la ratifica giunge in Senato *in extremis*. Allo stesso tempo rileviamo la presenza all'interno dell'Accordo di criticità che, se non adeguatamente monitorate, potrebbero portare verso l'insuccesso dell'intesa e tradursi anche in effetti negativi per il nostro Paese. Nella brevità di questa dichiarazione di voto riprendo rapidamente qualche punto. Innanzitutto, va evidenziata la cadenza delle verifiche che avranno periodicità di cinque anni, secondo quanto indicato nel Protocollo, all'articolo 4, punto 9). È vero che tutti i Paesi sottoscrittori hanno aderito a un unico sistema di verifica degli impegni presi, tuttavia ci pare che il periodo di cinque anni possa comportare deviazioni non conformi all'obiettivo finale (il primo impegno 2020, che è la verifica della prima applicazione, è fissato al 2023). L'accordo per il monitoraggio degli aggiornamenti sugli impegni assunti dagli Stati è quindi argomento molto delicato, da monitorare costantemente insieme all'aggiornamento del bilancio globale di cui all'articolo 14. Un'altra criticità che è necessario evidenziare è legata agli impegni di ciascun Paese in ambito europeo. Il nostro Paese ha già fatto tanto nel settore dell'efficienza e delle energie rinnovabili ed è pertanto necessario che in ambito europeo si definiscano regole ed obiettivi per ciascun Paese improntati all'equità citata all'articolo 4 del Protocollo. La partita è aperta: sollecitiamo in questo ambito la definizione di criteri adeguati e tali da non penalizzare il nostro Paese, i cittadini e le imprese. Riteniamo cioè che si debba lavorare affinché non si attribuiscano all'Italia obiettivi troppo gravosi a causa del mancato impegno di altri Paesi. Inoltre evidenziamo, quale presupposto per una operatività ordinata e produttiva dei risultati, la necessità di un urgente aggiornamento della Strategia energetica nazionale, dato che essa dovrà necessariamente integrarsi con gli impegni assunti in sede di COP21 e nel recepimento del pacchetto europeo per l'energia, fornendo finalmente un quadro di riferimento coerente e capace di definire chiare linee di sviluppo di questo vasto settore. L'incertezza, lamentata in più occasioni dagli operatori pubblici e privati del settore, non giova al perseguimento degli obiettivi e soprattutto non giova all'economia. «Efficienza» sembra proprio essere la parola più adatta, da mettere in campo con un'azione trasversale in tutte le attività economiche, pubbliche e private, italiane. Un ultimo punto. La ratifica del protocollo rappresenta per il nostro Paese un'importante opportunità per modernizzarsi ed aggiungere efficienza, un'opportunità per le tecnologie italiane, tra le migliori al mondo, di essere collocate a supporto dello sviluppo di altri Paesi. Questa è una questione che, a mio avviso, stiamo trascurando e per la quale c'è la necessità di un rafforzamento dell'impegno. Nel protocollo vediamo infatti una grande occasione per tutte le aziende italiane che si occupano di efficienza energetica, di produzione da fonti rinnovabili, di implementazione di nuove tecnologie, alla condizione che ci si collochi nella prospettiva di fornire adeguato supporto amministrativo e finanziario per l'internazionalizzazione. Dobbiamo porre in condizione le aziende di casa nostra, soprattutto le di arrivare attrezzate per operare sui mercati esteri. In tal senso, ho presentato un ordine del giorno, che è stato accolto e che mi auguro si traduca rapidamente in azioni concrete. Supportare questo tipo di aziende contiene un alto moltiplicatore per la crescita economica del nostro Paese. Nel settore, a livello globale, ci sono impegni per 100 miliardi di dollari al 2025, destinati ai Paesi in via di sviluppo. Su questi finanziamenti le nostre aziende possono e debbono cogliere le migliori opportunità collocando sul mercato mondiale prodotti, sistemi e metodiche di gestione frutto di competenza e capacità di innovazione. Alla luce di queste considerazioni e nella consapevolezza che il percorso di attuazione dell'Accordo di Parigi richiede il costante monitoraggio attivo delle potenziali criticità che esso può comportare, dichiaro il voto favorevole del Gruppo di Forza Italia.

al ministro Galletti, per avere fatto svolgere al nostro Paese soprattutto nella fase di preparazione di questo Accordo, che ricordo ai colleghi un po' smemorati si è costruito durante il semestre di Presidenza italiana dell'Unione europea, un ruolo da protagonista, che ha fatto sì che esso oggi possa essere ratificato. È un accordo storico, importante decisivo che entrerà in vigore il prossimo 5 novembre, e che nell'appuntamento di Marrakech di novembre avrà un primo, nuovo

come il sistema industriale stia già cambiando, perché tutti i Paesi europei sono già proiettati verso un'economia circolare a bassa emissione di carbonio, con investimenti in innovazione e nuova tecnologia che ci potranno consentire di raggiungere gli obiettivi

Ce lo ha ricordato, un po' di tempo fa, un moderno e incompreso politico, un ambientalista e scrittore del calibro di Alexander Langer ed è con le sue parole che vorrei concludere questa dichiarazione di voto, con la quale annuncio il voto favorevole del Gruppo Partito Democratico. Alexander Langer ci disse che «Se non si radica una concezione alternativa (...), e se non si cerca in quella prospettiva il nuovo benessere, nessun singolo provvedimento, per quanto razionale, sarà al riparo dall'essere ostinatamente osteggiato, eluso o semplicemente disatteso».

Signor Presidente, proprio ieri mattina, al termine dei lavori dell'Assemblea, il nostro collega Airola ha svolto un intervento di fine seduta nel quale denunciava l'asimmetria di informazione da parte dei quotidiani e delle televisioni a favore del sì al *referendum* che si terrà il 4 dicembre. Ha citato il presidente Napolitano, chiamandolo - come potete leggere sul Resoconto stenografico - «presidente emerito», mentre ha citato Obama senza precedere con alcun titolo il nome; eppure non solo è Presidente degli Stati Uniti, ma è anche premio Nobel. Pertanto, la locuzione pronunciata dal presidente Zanda, «si deve sciacquare la bocca», è davvero fuori luogo, non pertinente e, lasciatemelo dire, di pessimo gusto. Voglio anche stigmatizzare, sempre dal Resoconto stenografico, che a metà del discorso il collega Airola è stato oggetto di «Commenti dal Gruppo PD»; quindi appare evidente che, durante il suo discorso, anche il Gruppo PD ha rumoreggiato, come capita di sovente. Quindi non lo fa solo il che il giudizio espresso dal presidente Zanda nell'affermare che in Parlamento ci siano persone «senza meritare di esserci» sia davvero offensivo, non solo per i milioni di italiani che hanno votato il Movimento 5 Stelle, ma anche per l'Istituzione stessa. Io sono medico da ventinove anni e noto nelle parole del presidente Zanda, che purtroppo non è la prima volta che fa questo tipo di discorso, una certa preoccupazione, caratterizzata da un certo nervosismo tendente alla persecuzione. Posso capire le difficoltà di un Capogruppo di maggioranza, incapace anche oggi di sostenere il numero legale, tanto è vero che sono venuti in soccorso diversi Gruppi di opposizione o presunta tale,

definire volgare un intervento del collega Airola che di volgare proprio non ha nulla è, non solo per il Capogruppo del Movimento 5 Stelle, ma per tutti gli italiani che hanno votato il Movimento 5 Stelle, inaccettabile. Respingiamo le accuse al mittente. Presidente Zanda, stia sereno!

e porre all'attenzione dell'Assemblea un episodio che ha colpito la mia attenzione, ma - penso - anche la nostra sensibilità. Nonostante viviamo in un Paese in cui è stata conquistata la libertà di stampa, di pensiero e di parola in generale, ci sono Paesi al mondo in cui nel 2016 ancora si va in prigione per una frase di troppo, per un racconto mai neanche pubblicato. Questo è successo a Golrokh Ebrahimi Iraee, scrittrice iraniana, condannata a sei anni di carcere per il romanzo mai pubblicato che è stato rinvenuto nel suo *computer*. La pena è stata computata in sei anni di carcere, cinque anni per offese all'Islam e uno per propaganda anti-governativa. Ebbene, il racconto considerato offensivo dell'islam narrava la storia di una giovane iraniana che guarda in televisione il film «The Stoning of Soraya M», la vera storia di una connazionale uccisa a pietrate, e si indigna fino a bruciare una copia del corano. Infatti, in Iran la lapidazione è consentita dal codice penale in quanto ritenuta «effettiva nel prevenire i crimini e proteggere la moralità».

la solidarietà, la stima e l'incoraggiamento a non mollare. Allo stesso modo, il nostro sguardo premuroso e umanitario vada ad accarezzare il viso spaventato e innocente di Sharbat Bibi, la rifugiata afghana con gli occhi verdi resa famosa dal fotografo Steve McCurry. È stata imprigionata con il pretesto di aver falsificato il documento di identità computerizzato in Pakistan. Quest'anno in estate, nella città pugliese di Otranto, alle immagini di McCurry è stata dedicata una mostra visitata da migliaia di persone.

Presidente, intervengo per ricordare una persona che è mancata oggi e che ha segnato la storia della televisione italiana: Luciano Rispoli, una persona che molto di noi hanno conosciuto e che si è caratterizzata per la sua

un uomo di televisione a tutto tondo, una persona gentile, un vero signore, un uomo che ha sempre servito la televisione senza servirsene come, a volte, molti fanno ricercando l'*audience* a qualunque costo. Rispoli ha rispettato gli altri; ha rispettato soprattutto il nostro Paese. È stato un italiano di cui essere orgogliosi e per questo io, che ho avuto il privilegio di conoscerlo, volevo ricordarlo solennemente in questa Aula del Senato.

condividere le sue valutazioni sulla serenità, la competenza, l'equilibrio, la cultura e l'amore per l'Italia. Penso che la Presidenza del Senato farà pervenire a nome di tutti un messaggio di cordoglio ai familiari di Luciano Rispoli.

di fatto si riconosce che, al di là delle gravi accuse che vengono mosse alla magistrata, non si può dimenticare che la stessa ha fatto in modo che molti beni

oltre a usare queste macchine blindate sottoforma di taxi, la signora Saguto ha anche utilizzato i poliziotti della scorta per farsi fare dei servizi personali.

anche in una posizione di debolezza in quanto la magistrata ovviamente conosce bene il prefetto, è superiore ai poliziotti stessi, ragion per cui devono derogare a ciò che non dovrebbero fare e lo fanno. Il punto, quindi, è sempre lo stesso, ovvero se sia necessario dare la scorta a certi soggetti,

Il 6 agosto del 2014 chiedemmo, con un'interrogazione al Ministro dello sviluppo economico, se non ci fossero rischi e conseguenze per l'economia e la politica italiana sulla svendita di *asset* di interesse strategico nazionale alla società cinese State grid international development. Ci riferivamo alla cessione

Allora eravamo preoccupati e chiedemmo quali conseguenze l'accordo avrebbe avuto in Grecia, dove China Grid partecipa come concorrente di Terna all'acquisizione della quota di maggioranza del gestore della rete elettrica ellenica, con il manifestarsi della situazione dove controllante e controllata competono per lo stesso obbiettivo; e se la strategia complessiva di penetrazione nell'area mediterranea da parte cinese fosse stata effettivamente valutata. valutata. Il Governo ci rispose di stare tranquilli, talmente tranquilli che, a pensar male, ci abbiamo azzeccato. Infatti, è notizia sui quotidiani di oggi che i cinesi sorpassano Terna nella corsa all'acquisto dell'*utility* greca. Il colosso cinese State Grid ha presentato, cioè, l'offerta più alta e si è aggiudicato il 24 per cento della *utility* greca. Questo era in concorrenza con Terna che, insieme al fondo F2i, aveva presentato un'altra offerta la scorsa settimana. Quindi abbiamo perso! Un risultato molto negativo per il Governo Renzi in un settore chiave e strategico di politica nazionale ed estera, ormai ceduta al soldo cinese. Probabilmente tale risultato avrebbe fatto rabbrividire perfino Enrico Mattei che credeva utile per l'Italia il raggiungimento di un'autonomia politica praticabile solamente se capaci di avere un'autonomia energetica dall'estero. Al momento, prendiamo atto che questo Parlamento e questo Governo vanno nella direzione contraria. Ah! Naturalmente, è tutta colpa della Costituzione!

nell'ambito di una commemorazione (così venne definita a posteriori) per un fatto accaduto a Fermo: censura preventiva. Sono poi andato a controllare e ho visto che solo al tempo del fascismo era capitato che in Parlamento venisse tolta la parola a un parlamentare prima ancora che potesse esprimere il suo pensiero. Di questo episodio, che considero gravissimo, ho immediatamente informato, tramite lettera, il Presidente del Senato perché prendesse posizione, a maggior ragione quando la commemorazione

raccontate. Per mesi - luglio, agosto, settembre e ottobre - ho atteso una risposta da parte della Presidenza del Senato, che ieri finalmente mi è arrivata. Ne do lettura perché credo riguardi tutti i colleghi: «Onorevole senatore, la informo di aver trasmesso dice il Presidente del Senato - alla vice presidente Lanzillotta, per opportuna conoscenza, copia della lettera e annessa documentazione da lei inviatemi in relazione a una parte della seduta antimeridiana dell'Assemblea del 7 luglio, presieduta dalla stessa senatrice».

Si decide, quindi, di abbattere questo albero. La patologia che colpisce gli ulivi è sempre quella famosa sputacchina che, in questo caso, avrebbe percorso chilometri e chilometri per posarsi, ripeto, su un solo albero di ulivo.

ciò è veramente ridicolo, ma è davvero assurdo che la *xylella* si possa propagare attraverso qualcosa, a meno che non ci sia la manina dell'uomo che ne conduce

queste le problematiche da affrontare. Bisogna continuare a vigilare e soprattutto impedire che la solita mano dell'uomo continui a desertificare quelle terre, che sono ricche e vogliono continuare a produrre. stesse terre martoriate dalla volontà dell'uomo e - soprattutto - di questo Governo che continua a mercificare e scambiare i nostri prodotti con la fetecchia del mondo internazionale.